Presidente, vorrei sottolineare come anche negli ultimi giorni si siano verificati ripetuti e gravi infortuni,

restanti che non sono stati dichiarati improponibili è contrario sulla base dei ragionamenti che sono stati sviluppati ieri. In primo luogo, si tratta di mantenere il testo che è stato approvato alla Camera in modo da poter approvare la legge in tempi

di mantenere questa, che è stata frutto anche di un accordo alla Camera; quelle proposte sono delle formule anche interessanti, che si ispirano, ad esempio, al modello delle elezioni politiche spagnole, ma si ritiene preferibile la forma contenuta nel disegno di legge così come è stato approvato dalla Camera. Vi sono poi delle proposte per fronte al problema del cosiddetto slittamento dei seggi. Già erano state avanzate nel 2004: si tratta, ad esempio, di proposte per introdurre un

poter necessariamente essere manifestate in un'Aula parlamentare, men che meno del Parlamento europeo. Vi sono diverse

È interessante anche notare che in altri Paesi vi sono forme di sbarramento implicite assai più alte; e non credo proprio che possiamo ritenere che, ad esempio, la Francia

rappresentanze di pochi partiti, senza frammentazioni inutili, che danno certamente un diritto di tribuna ad alcune formazioni, le quali però poi di solito non si riconoscono in alcuno dei grandi partiti europei e dunque incontrano grandi difficoltà ad apportare il loro contributo al lavoro parlamentare. Pertanto, ribadisco il parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

sicuramente costituiranno il contenuto di un provvedimento organico che affronterà complessivamente la materia.

che gli eletti venissero sempre dalla Sicilia proprio per la dimensione demografica di quest'isola. già nel prossimo Consiglio dei ministri il Governo intende portare un provvedimento *ad hoc* che consenta lo scorporo della Sardegna dalla circoscrizione Sicilia-Sardegna,

così com'è stato rappresentato ieri da senatori sia di maggioranza sia di opposizione. In quella sede porteremo questo provvedimento e daremo una risposta anche a questo tema.

senatore Malan credo abbiano confermato quale sia in effetti il problema qui dentro; la violazione dei diritti civili e politici porterebbe via almeno due giorni di dibattito, ma in merito alla proposta di modifica dal sistema elettorale, fatta in corso d'opera a due mesi e mezzo dalla chiusura delle liste, chiaramente essa va nella direzione a mio avviso opposta alla possibilità per i cittadini italiani di partecipare in maniera paritaria a questo tipo di tornata elettorale. Il problema non è la dimensione del partito né tanto meno la frammentazione. Se aveste ridisegnato i collegi ‑ e grazie alle tecniche esistenti sarebbe stato possibile farlo nel giro di una settimana, o della nottata in cui vi siete messi d'accordo per modificare questa legge elettorale ‑ facendone 72, la Sardegna, visto e considerato che anche il ministro Calderoli ne ha parlato fino or ora, avrebbe potuto esprimere finalmente un eurodeputato.

Denuncio anche il fatto che non si vuole mettere agli atti chi è a favore di questo tipo di provvedimento, sia non sostenendo il voto elettronico, sia,

dovesse infastidire i miei colleghi. Comprendo le ragioni della grande maggioranza del Parlamento che vuole concludere velocemente questo *iter* legislativo

ore qualcuno che è stato semplificato e che è stato particolarmente impegnato nel definire questo assetto legislativo.

anche forze politiche che hanno un loro radicamento culturale, e mi riferisco alle esperienze sia di estrema sinistra che di estrema destra. In particolare, soprattutto

il sistema elettorale precedente che ha garantito al Parlamento europeo una rappresentanza ricca e variegata che, comunque, per la grandissima parte - mi spiace contraddire il relatore Malan - è poi confluita nelle grandi famiglie del non determinando alcuna frammentazione. È un'altra, infatti, la funzione politica del Parlamento europeo: è una tribuna di opinioni che tentano di costruire una cultura istituzionale europea e non è un'assemblea un'assemblea che deve garantire governabilità ad un qualsiasi governo. Questo atto politico per ragioni puramente interne restringe fortemente - e non dico

Presidente, prima ho sbagliato il riferimento all'emendamento: il voto era favorevole e infatti ho pigiato il tasto verde. Anzi, ringrazio il senatore Pistorio per la sua opera di cesello, nel tentativo di riportare il sistema elettorale che ha mandato gli eurodeputati nel 2004

mediazione tra l'auspicata esigenza di semplificazione del quadro politico che questa legge *bipartisan* determina, *bipartisan* determina, e l'opportunità di consentire a forze politiche significative dell'esperienza culturale italiana di essere presenti nel Parlamento europeo. Esso individua una soglia mediana, signora Presidente: non più il 4 per cento, che è una soglia oggettivamente elevata e che mal si concilia con le ragioni che le elezioni europee dovrebbero assistere in termini di rappresentanza politica, ma una soglia più bassa e politicamente che non mortifica e non taglia le gambe a tante esperienze politiche. Tra l'altro, questa soglia è perfettamente coerente. Infatti, poiché miei colleghi di miei colleghi di ambedue gli schieramenti mi hanno ricordato come il 4 per cento sia la soglia di sbarramento prevista per le elezioni politiche nel nostro Paese e si è quindi semplicemente riconfermato quel tipo di

accettando l'ipotesi di uno sbarramento significativo ma non ostativo, vorrei richiamare a un minimo di coerenza proponendo una soglia del 2

ma lo illustrerò successivamente - una doppia soglia nel caso di tipo circoscrizionale, che avrebbe il senso di consentire la rappresentanza ai partiti territoriali. Credo che in questo Parlamento vi siano alcune esperienze territoriali molto forti che non dovrebbero perdere la memoria di quello che sono stati prima di diventare un grande partito nazionale e dovrebbero consentire che si determinino le condizioni per l'affermazione di partiti territoriali, se vogliamo un federalismo bilanciato geograficamente. in dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo, anche a nome della senatrice Poretti. Non mi convince il ragionamento del senatore Pistorio, che sembra essere fatto piuttosto *ad hoc* per alcuni partiti a presenza regionale, anche se non se non ha tutti i torti su quanto ha testé ricordato in merito alla coalizionabilità di forze politiche che già esiste relativamente alla legge elettorale nazionale. Non mi convince in particolare l'esordio del suo ragionamento.

che si è messa d'accordo nelle segrete stanze per avere un sistema elettorale che loro sperano porti qualcuno dei loro attivissimi eurodeputati a Bruxelles o a Strasburgo; ci asterremo, quindi, su questo emendamento.

Presidente, colleghi, l'emendamento 1.122 è l'ultimo tentativo. Voglio dare ragione al collega Perduca: è vero, in questi emendamenti c'è anche il tentativo di preservare o, meglio, consolidare un'esperienza territoriale e, quindi, hanno una *ratio*. A noi andava benissimo la legge esistente; vorremmo una soglia più bassa di tipo nazionale, ma saremmo disponibili - e lo dimostreremo impegnandoci nelle elezioni, perché noi non ci facciamo semplificare e quindi concorreremo con il nostro simbolo - anche ad accettare lo sbarramento del 4 per cento, se però ci fosse anche una coerenza di sistema. So che non basterebbe il voto degli amici della Lega, abbiamo tante volte ragionato di meccanismi elettorali ed istituzionali che debbono consentire, se non incoraggiare, le esperienze

l'altro con qualche crepa forse comincia a sviluppare qualche riflessione al suo interno rispetto a processi di unificazione che mi paiono complicati. Questo è, comunque, un problema che non mi riguarda un Paese che sceglie la strada federalista e della rappresentanza degli interessi dei territori e deprime le rappresentanze politiche che assumono il territorio come riferimento originale ed esclusivo ed esclusivo degli interessi che intendono rappresentare. Prevedere una soglia di sbarramento circoscrizionale doppia rispetto alla soglia nazionale vuol dire

cento è un valore assolutamente rilevante politicamente, che però costituisce il riconoscimento dell'esperienza politica dei partiti territoriali. Ministro Calderoli, lei mi ha sempre ricordato che ci sarebbe una direttiva europea che impedisce la doppia soglia: non mi risulta; è un'interpretazione un po' forzata che rispetto anche per la sua ormai grande perizia istituzionale, ma ricordo a lei, all'uomo che ha lavorato tanto per l'affermazione dei principi federalisti e dei partiti territoriali, che questa clausola sarebbe il riconoscimento politico e istituzionale di un'interpretazione della nostra storia politica che oggi tende al modello

che tendono alla semplificazione del quadro politico, e forze che invece vogliono rimanere legate al territorio per garantirne gli interessi e rappresentarne le vocazioni più autentiche. Per questa ragione, sono convinto che l'emendamento 1.122 poteva essere un punto di intesa ragionevole, se soltanto non vi fosse stata questa blindatura inaccettabile del Parlamento, definita fuori di esso dai vertici di un sistema politico che oggi, almeno per una parte, entra in crisi.

il cui contenuto mi convince molto più di quello presentato precedentemente. In effetti, il raggiungimento dell'8 per cento in un collegio regionale va nella direzione auspicata dagli estensori di questa modifica del sistema elettorale, perché chiaramente un partito che arriva a raccogliere tanti voti quanti sono i cittadini di almeno dieci Stati membri dell'Unione europea - non dico messi insieme, ma presi uno per uno - sicuramente merita di avere rappresentanti in Parlamento. Faccio mie tutte le considerazioni e non però, come sentite, la passione del senatore Pistorio, salvo la fiducia nella possibilità di vedere un *moloch* smottare e avere un effetto domino anche nei confronti dell'altro: la fiducia va nutrita quotidianamente di lotta politica. Comunque, per questo il nostro voto è a favore e chiediamo

Presidente, ringrazio il senatore Perduca non soltanto per la condivisione parlamentare della battaglia di questa mattina, ma anche per aver offerto un ragionamento

rivolgo agli amici della Lega Nord, che oggi navigano con numeri molto più ampi, ma che non avevano meno ragione nella loro azione politica quando stavano al 3,9 che al 3,9 per cento sarebbero rimasti fuori dal Parlamento europeo: questa norma non avrebbe loro consentito di interpretare le giuste istanze dei territori che essi rappresentano in modo assolutamente rispettoso di quell'azione politica. Tra il 3,9 e il 4 per cento non vi è una differenza di qualità democratica o di capacità politica. Tante ragioni possono determinare un esito elettorale e la Lega non era meno impegnata sul territorio quando stava al 3,9 per cento e non era tanto tempo fa.

perché è ingiusto impedire ai partiti territoriali di esprimersi in termini di rappresentanza istituzionale. A volte ci sono gesti simbolici che non producono un effetto concreto, ma che saldano una sintonia culturale e politica.

nella direzione contraria da quella da voi auspicata circa le frammentazioni, perché si creeranno cartelli elettorali che il giorno dopo le elezioni si ridivideranno un'altra volta all'interno del Parlamento.

essere favorevole ad uno sbarramento territoriale. Il problema è che stiamo dando esecuzione ad una direttiva europea che parla di soglia e non di soglie; quindi è evidente che la soglia può essere solo

Signor Ministro, vi sono state occasioni in cui è stato più brillante. Questa disquisizione tra soglia e soglie, come impeditiva, francamente non è da ministro Calderoli come lo conosco e lo apprezzo.

Questa legge non ha consentito di affrontare in modo organico i problemi e quindi modificare le circoscrizioni ed i meccanismi elettorali. Ci avete messo di fronte ad una bevanda preconfezionata: o bere o affogare. E qui stiamo affogando noi!

fare una dichiarazione di voto, anche a nome delle senatrici Poretti e Bonino, a favore di questo emendamento. Si vede, caro collega, che la semplificazione passa anche attraverso la discriminazione nei confronti dei miopi. Il Governo ha da poco ratificato la Convenzione internazionale per i diritti dei disabili e si rifiuta di allargare di 10 millimetri - pensate voi!

una risorsa e un'opportunità per incoraggiare meccanismi di aggregazione, che ovviamente passano anche dal riconoscimento del simbolo. Se voi avete intenzione di semplificare ma non di impedire una competizione ed una proposta chiara, un simbolo leggermente più grande può consentire a forze politiche diverse di apparentarsi e di trovare delle soluzioni organizzative e politiche coincidenti, mantenendo la loro riconoscibilità presso

questo il diniego su questo emendamento è la conferma di una scelta drastica, troppo drastica, che mal si concilia con la natura delle elezioni europee.

Sono certo di interpretare l'animo di tutti i colleghi nel rivolgere un convinto ringraziamento alle forze dell'ordine per per l'arresto, operato questa notte, dei due presunti autori della terribile violenza avvenuta a Roma nei giorni scorsi contro una ragazza

indagini pronte e risolutive, una giustizia severa ed efficace, una pena che corrisponda alla gravità dei reati e che sia scontata nella sua pienezza. Con convinzione rinnovo oggi, a nome di tutta l'Assemblea, la solidarietà e la vicinanza a tutti coloro che sono vittime di violenze atroci ed ingiustificate, qualunque sia la loro nazionalità o la loro etnia. Ricordo che nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di esprimere questi sentimenti anche nei riguardi di un cittadino indiano oggetto di un'insensata e crudele aggressione da parte di nostri connazionali, anch'essi identificati dalle forze dell'ordine. La nostra solidarietà va a tutti coloro che hanno sofferto e la nostra condanna è per gli autori di questi reati, qualunque sia la loro nazionalità.

Signor Presidente, signori membri del Governo, a nome della delegazione delle Autonomie e della Südtiroler Volkspartei, esprimo voto decisamente negativo a questa modificazione della legge n. 18 del 1979. Questo accordo tra grandi partiti è solo un accordo di convenienze e di potere che non permette la rappresentatività di piccole realtà e di specificità come quella valdostana e dell'Alto Adige, peraltro - lo sottolineo - riconosciute dalla Costituzione. In particolare, la legge, non modificata come avevamo richiesto noi, obbliga le minoranze linguistiche riconosciute ad apparentamenti non sempre naturali; per la Valle d'Aosta, nello specifico, la soglia dell'apparentamento a 50.000 voti ha sempre precluso, tranne che in un caso, l'elezione di un parlamentare europeo valdostano.

In un'Aula come questa, signor Ministro, in cui si è appena parlato di federalismo, ora ritorna invece la legge dei grandi numeri, che esclude chi i grandi numeri non li ha e non li può avere. Questo provvedimento smentisce, infine, le promesse fatte da *leader* di grandi partiti nazionali, che chiudendo la campagna elettorale per le elezioni politiche in Val d'Aosta avevano promesso un candidato valdostano alle elezioni Termino dicendo che tutti parlano di rispetto delle autonomie, ma il disegno di legge in esame in pratica le mortifica pesantemente. Signor Presidente, colleghi, è in piena armonia con l'intervento del collega Fosson che formulo quest'ultimo intervento su una materia, che ha visto un'intesa da

che l'intesa è stata definita su un punto di equilibrio che ha accordato le esigenze non soltanto dei partiti grandi ma anche di quelli medi, ma tutti caratterizzati per essere partiti nazionali, che difendono il loro ruolo di partiti nazionali e che hanno fatto strame in questo caso della cultura delle autonomie che la nostra Costituzione riconosce e che ha sempre trovato, anche nelle norme elettorali, accorgimenti per non mortificare questa esperienza. in discussione vengono mortificate grandi tradizioni culturali che forse il nostro Paese considera ormai desuete, anticaglie della storia, che devono essere chiuse in uno sgabuzzino. Penso alle tradizioni repubblicane, socialiste, liberali, ma anche alla novità che sta emergendo in piena sintonia non soltanto con la nostra Costituzione formale, ma con quella che sta divenendo la Costituzione materiale del nostro Paese. Un Paese che - ricordo - riconosceva il valore delle autonomie, delle minoranze linguistiche, che riconosceva le autonomie anche di Regioni importanti come quelle a Statuto speciale determinate da condizioni particolari della loro storia civile e che sembrava avere scelto, con la riforma di tipo federalista, la valorizzazione delle autonomie come sistema per garantire un avanzamento della nostra convivenza civile, dell'efficienza della nostra pubblica amministrazione, della volontà di riunificare concretamente questo Stato in cui il modello centralista ha miseramente fallito. Ma ricordate che non ci può essere federalismo, non ci può essere uno Stato che riconosce le autonomie se non viene salvaguardata l'esperienza dei partiti autonomistici. Signor Presidente,richiamando la sua attenzione, voglio

che ha goduto in termini formali di grandi prerogative derivanti dallo Statuto speciale antecedente alla Carta costituzionale e che è parte integrante di quella stessa Carta, la classe la classe dirigente - non quella attuale, che si misura con un'altra esperienza - ha tradito le grandi aspettative del Sud autonomistico non coltivando questo valore e asservendo la sua azione politica alle indicazioni del potere centrale. Il tradimento autonomistico consumato in Sicilia è il frutto di una classe dirigente che non ha coniugato la scrittura costituzionale con la concreta azione politica. Il Movimento per l'autonomia, che è nato in Sicilia e che intende diffondere questi principi in tutto il Paese e in particolare al Sud, ritiene che vi debba essere una nuova stagione delle autonomie. Se lo Stato

non dico favorire ed incoraggiare questo aspetto, ma almeno riconoscerlo. Non si possono disgiungere gli aspetti costituzionali da quelli elettorali. Occorrono forze politiche autonomiste per dare sostanza all'autonomia. al tema delle elezioni europee e quindi elezioni che non devono definire maggioranze di governo o un'Assemblea chiamata a sostenere un Esecutivo, ma semplicemente garantire rappresentanza ad esperienze politiche e a territori, è la legge peggiore in cui introdurre questo meccanismo di blindatura, che anche la concreta azione parlamentare ha definito con

legge in esame contraddice totalmente la sostanza del processo politico italiano per come viene enunciato, perché mortifica le esperienze identitarie e quelle territoriali. Siccome siamo convinti delle nostre buone ragioni

Non ci faremo impaurire e affermeremo le ragioni legate al valore dei territori, alle loro esperienze e ai loro interessi, ma anche più concretamente al valore dell'autonomia,

perché queste elezioni, anche grazie al nostro contributo, possano offrire a tante esperienze politiche e territoriali un luogo di cittadinanza, una sede in cui misurarsi con gli elettori, perché di queste voci originali non sia privato il nostro panorama politico e perché al Parlamento europeo possa sedere una rappresentanza più diffusa degli interessi, delle culture e dei territori italiani, perché non credo bastino due partiti a rappresentare la dialettica politica del nostro Paese. Presidente, colleghi, intervengo brevemente per puntualizzare alcuni passaggi. L'Italia dei Valori ha dato

Innanzitutto, l'Italia dei Valori si è sempre misurata con soglie di sbarramento e nel 2001, pur non avendo raggiunto

oggi può con tranquillità affrontare uno sbarramento che nel 2001 non ci permise di entrare in Parlamento. La semplificazione è un processo a nostro avviso non più arrestabile. La semplificazione non significa creare due calderoni indistinti, ma significa riuscire a creare all'interno del Parlamento italiano - anche all'interno del Parlamento europeo rappresentanze italiane che poi si riconoscano nelle grandi famiglie europee. Per questa ragione, il Gruppo dell'Italia dei Valori, che pure avrebbe voluto una soglia di sbarramento più contenuta, per non dare alcuna impressione di una compressione della partecipazione di di associazioni, di organismi, di partiti, di movimenti che pure sono sul territorio, accetta questa sfida e auspica

di mettere insieme, non un cartello elettorale, ma un cartello culturale e quindi elettorale, per affrontare e superare la soglia di sbarramento. Colleghi, questa è una soglia di sbarramento che - implicita o esplicita - è nelle più grandi democrazie europee:

dell'Italia dei Valori è convinto che non avere introdotto liste bloccate sia una conquista per tutti;

dà la possibilità al cittadino elettore di conoscere, scegliere, votare anche le persone e non solo i partiti politici. Per queste ragioni, il Gruppo dell'Italia dei Valori darà il suo voto favorevole a questo disegno di legge. Signor Presidente, il voto della Lega Nord Padania è favorevole alla razionalizzazione della rappresentanza politica dei cittadini, e la riduzione della frammentazione è un requisito fondamentale affinché i partiti possano svolgere quel ruolo di sintesi che la Costituzione attribuisce loro, quel ruolo di cerniera tra i cittadini e questo Stato che deve essere sempre più riformato: siamo, in questo senso, sulla buona strada. Credo che qui non si voglia nascondere nulla o mettere nulla nel ripostiglio, caro senatore Pistorio, cari amici del Movimento per l'autonomia: non dobbiamo confondere l'identità e l'autonomia con lo spreco, con il ricatto, con l'auto-conservazione del partito; è semplicemente questo il nostro pensiero. La Lega Nord ha affrontato la questione di democrazia posta dalla soglia di sbarramento fissata al 4 per cento e, come ho già avuto modo di dire in discussione generale, questa soglia, a nostro parere, costituisce invece un modo superiore di adempiere alla più larga e manifesta volontà popolare.

Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo a votare e per il quale preannuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Partito Democratico non costituisce certamente una riforma elettorale organica. signor Presidente, vorrei ribadire qui, a nome del mio Gruppo, l'assoluta necessità di mettere mano in modo serio e ordinato alla delicata vicenda della materia elettorale. Non è immaginabile, non è consentito e non è coerente che in Italia si abbia cinque diversi sistemi elettorali a seconda del livello territoriale con cui si procede alle elezioni. Avvertiamo l'esigenza di un sistema elettorale certamente caratterizzato per ognuno dei livelli, ma con un'impostazione di fondo sostanzialmente coerente. Voglio anche aggiungere che il disegno di legge che ci accingiamo a votare non risolve neanche tutte le questioni emerse con grande chiarezza nel corso del dibattito ed esposte in quest'Aula, in particolare dai relatori.

Nel momento in cui l'Europa è sempre di più delle Regioni e delle comunità locali, avvertiamo l'esigenza che i nostri rappresentanti nel Parlamento europeo abbiano un rapporto diretto di conoscenza - e di essere riconosciuti - con il territorio che rappresentano. è un'altra esigenza, ossia quella di risolvere la questione ormai troppo lunga della Sardegna, una grande Regione di questo Paese che sistematicamente non ha eletti nel Parlamento europeo. Mi permetto di ricordare che l'isola di Malta, in virtù del fatto che è uno Stato, ha se non ricordo male tre rappresentanti nel Parlamento europeo, pur avendo un quarto o un quinto della popolazione dell'isola della Sardegna. è un'ulteriore questione da risolvere e mi rivolgo in particolare a lei, signor Presidente, che tra l'altro è della mia terra, la Sicilia: in virtù di questo aberrante sistema di attribuzione dei seggi all'interno dei singoli partiti, accade che le circoscrizioni minori, in particolare quella delle isole, sistematicamente eleggano molti meno parlamentari di quelli a cui avrebbero diritto e regalino i propri rappresentanti ad altre circoscrizioni molto più ampie. Paradossalmente, Regioni come la Sicilia e la Sardegna o le circoscrizioni minori, che avrebbero bisogno di avere una forte voce a Bruxelles, non ce l'hanno a causa di un sistema elettorale che, da questo punto di vista,

femminile nel Parlamento europeo. La presenza italiana è al di sotto della media europea equesto è assolutamente intollerabile*.

abbiamo raggiunto l'intesa tra tutti i Gruppi affinché, subito dopo le elezioni europee, si riprenda l'esame della legge elettorale anche per il Parlamento europeo, con l'impegno a risolvere le questioni che ho qui ricordato, che sono largamente condivise.

tutte - ovvero 26 forze politiche. Ma che razza di democrazia è un Paese in cui la presenza politica e parlamentare è sbriciolata in 26 forze politiche rappresentate in Parlamento?

rappresentanti di cinque, sei, forse sette forze politiche, sostanzialmente in media con tutti gli altri grandi Paesi dell'Europa. sia una riforma molto parziale, certamente produce un effetto positivo: quello di consentire una gamma di rappresentanza nel Parlamento europeo estremamente diversificata, da forze di destra a forze di sinistra passando per le forze di centrodestra e centrosinistra, ma nello stesso tempo una presenza non parcellizzata in un modo francamente inaccettabile. Ecco la ragione per la quale siamo convintamente favorevoli a votare questo provvedimento. Inoltre, rivendichiamo anche alla determinazione e all'impegno del Partito Democratico se oggi il testo che votiamo prevede il mantenimento nel sistema elettorale

Signor Presidente, colleghi senatori, diciamo subito che questa era l'unica modifica e l'unica intorno alla quale è stato possibile raggiungere un accordo. Lo ha ricordato ieri all'inizio del dibattito il senatore Ceccanti, tornando indietro nel tempo, ha sottolineato che questo accordo, raggiunto non senza fatica, poteva essere paragonabile a quello del 1995 sulla allora riforma della legge elettorale per le elezioni regionali. Io fui al centro e artefice di quell'accordo, che non credo si possa sminuire rispetto al disegno di legge che stiamo approvando oggi. Voglio ricordare a me stesso che nel 1995 il Paese viveva un momento di grandissima difficoltà: vi era vi era il Governo Dini, frutto di un ribaltamento dei risultati elettorali, vi era l'imminenza delle scadenze elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali in 15 Regioni a Statuto ordinario. Si mise mano ad una riforma, perché nel frattempo era intervenuta la modifica della legge elettorale, per via referendaria e non per accordo tra le parti politiche; quindi c'era la necessità di adeguare il sistema elettorale delle Regioni a quello che già si era determinato a livello nazionale. Facemmo un grande miracolo di mediazione, affidato all'indimenticabile Pinuccio Tatarella, relatore alla Camera, che introdusse in maniera artificiosa l'elezione diretta del Presidente della Regione, laddove in Costituzione tale indicazione non era prevista. Quindi, non si può paragonare il *maquillage* che facciamo oggi ad un accordo che nel 1995 aveva altro tenore ed era molto più esteso perché comunque rafforzava la nascita della democrazia bipolare e della democrazia dell'alternanza nel nostro Paese. Oggi siamo stati costretti ad un'intesa minimale. Introduciamo unicamente una soglia di sbarramento, quasi come se questo disegno di legge non fosse altro che il recepimento di una direttiva europea. Ci limitiamo a questo. Volevamo fare di più. Abbiamo tentato di fare di più, cercando di giungere ad un accordo più ampio. Ci sono stati fuochi di sbarramento; c'è stata indisponibilità diffusa. Gli ultimi mesi testimoniano chi non ha voluto un confronto più ampio, chi non ha voluto perseguire la strada di un'intesa più estesa. Pertanto, le riflessioni che hanno fatto in molti, da ultimo il senatore Bianco, sottolineano la necessità che sulle dinamiche e sui modelli elettorali il Parlamento si deve attardare perché molte sono le questioni aperte, innanzitutto la omogeneità dei sistemi elettorali. Ricordava il senatore Bianco che esistono cinque sistemi elettorali diversi per cinque livelli di attribuzioni della responsabilità di governo dei territori.

operato a sinistra dal PD e nel centrodestra dal PdL, due grandi partiti nazionali, sta a significare che la politica vuole semplificare, ma per farlo c'è bisogno che le regole che accompagnano l'attribuzione della responsabilità di governo

elettorali indicano questo) del sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Regione, ma poi molti sono contrari alle elezioni dirette del *Premier* e del Presidente della Repubblica. Non si capisce perché la democrazia diretta funziona quando si tratta di eleggere il sindaco o il Presidente della Regione ma non potrebbe funzionare se si dovesse eleggere il candidato *premier* o il Presidente della Molti si fanno offuscare da questioni personali e non guardano al sistema nella sua omogeneità e nella sua complessità. Allo stesso modo, alla questione che riguarda la rappresentanza e il legame con il territorio si può ovviare in tanti modi: lo

Si fa chiarezza su norme introdotte ad altri livelli. Ricordo le elezioni politiche e quelle regionali, laddove la nostra legislazione assegna rimborsi elettorali anche a forze politiche i cui candidati non risultano eletti. La questione di fondo è quella di chiarire se

e, quindi, permanendo l'equivoco, chiunque può leggere le questioni e le norme in maniera diversa, come è accaduto anche in questo nostro dibattito. L'altra questione aperta la presenza delle donne nella percentuale degli eletti. Si tratta di un problema di pari opportunità che questa legge tutela perché obbliga i partiti a candidare un numero di donne poi la questione delle elezioni. Molto spesso mi domando - ma è una domanda che non impegna gli altri - se la pari opportunità significa mettere nelle stesse condizioni di competitività uomo e donna oppure significa mettere in moto meccanismi che danno più opportunità ad un sesso rispetto all'altro. Anche di questo si dovrà parlare. però una questione di fondo che induce una riflessione sulla necessità che le regole imporranno, se vogliamo portarle fino in fondo e se vogliamo fare un confronto serrato e serio, anche alla determinazione che bisognerà modificare la nostra Costituzione. Oggi,

La Campania e la Lombardia, che pure hanno popolazioni estremamente più vaste, ne eleggono di meno: non c'è omogeneità neanche nel rapporto tra la popolazione e gli eletti. Non c'è omogeneità di legge elettorale a quel livello, perché ogni Regione si può fare la sua legge elettorale; ogni Regione può decidere il numero dei consiglieri regionali; ogni Regione può decidere persino la sua norma sulla ineleggibilità

anche di ritoccare la Costituzione. Nessuno può dire che si difende tutto a prescindere. Se un confronto deve essere serio fino in fondo, dobbiamo riprendere tali questioni e avviare un confronto di merito sereno e certo.

delle forze politiche nel corso delle ultime elezioni politiche (la norma elettorale infatti con atteggiamenti diversi avrebbe continuato a favorire la frammentazione). In questo caso, introducendo un

particolare quelle dei due colleghi dei due Gruppi più grandi, il Partito Democratico e il Popolo della Libertà. In entrambi le dichiarazioni, al di là del fatto che era acclarato ormai il voto favorevole, c'è stata un'elencazione di punti negativi della legge elettorale che non sono stati né presi in considerazione né risolti. Si dice che verranno presi in considerazione domani per essere risolti. Intanto abbiamo proceduto a questo atto, ossia a modificare la legge elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, alzando lo sbarramento al 4 Vorrei ricordare a tutti in quest'Aula che l'elezione dei membri del Parlamento europeo si basa su un principio di rappresentatività proporzionale e che è certamente lecito e possibile, così come recita la norma, applicare una soglia di sbarramento. elettorale si fosse fatto un ragionamento serio nei tempi dovuti e non a ridosso delle elezioni, a due mesi e poco più dalla presentazione delle liste e quindi a giochi già iniziati, a giochi già iniziati, avremmo tutti concorso per avere un risultato qualificato e certamente comprensivo di tutte le difficoltà che qui sono state evidenziate. Così non è stato. La fretta, che è sempre cattiva consigliera, e non solo la fretta, ma anche interessi che probabilmente qui sono poco visibili, ma che ci sono da ambo le parti, ha consentito questo colpo di mano, lo sbarramento al 4 per cento, che di fatto elimina la possibilità di espressione di forze culturali e politiche che in questo Paese hanno fatto molto per la democrazia. Esse vengono eliminate dalla possibilità di essere presenti a livello di Parlamento europeo, là dove contano le culture politiche che hanno

non è scaturito da un confronto serio né a livello parlamentare né del Paese, e sottende ad interessi, che non voglio qui elencare, di cui si vedono gli effetti negativi. I repubblicani europei, pertanto, anche perché portatori di una pedagogia civile che affonda le sue radici nei valori che sottostanno alla legalità repubblicana, voteranno decisamente contro.

Prego, senatore.

se era sbagliato anni fa dire che una legge elettorale non si fa a ridosso delle elezioni è sbagliato anche se il consenso è maggiore di allora. La seconda ragione è la questione della rappresentanza femminile e di genere, come hanno sostenuto peraltro, anche i relatori di maggioranza. una cosa che non per colpa sua non si è realizzata. Mi riferisco al patto di consultazione e al diritto di tribuna. Ora, non si fa una legge che esclude una parte senza nemmeno consultare questa parte; bisognava avere la la sensibilità istituzionale che lei aveva mostrato anche rispetto a questo problema. Questa astensione è anche un messaggio di non

ma di quale regole state parlando? Quelle fatte a partita iniziata per fare fuori i contendenti? Si è parlato di sbarramenti per la governabilità; di cosa, dell'Europa? Peccato che il Parlamento europeo non sia il Governo europeo, ha un ruolo politico più che legislativo, almeno finora. Le regole si cambiano, ma soprattutto si rispettano. Abbiamo visto elezioni elettorali regionali e locali senza tribune elettorali e senza regole televisive; abbiamo dieci anni di provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui si certifica la cancellazione, per esempio, dei radicali operata attraverso e per tramite della televisione di Stato. Senza conoscere non è dato deliberare.

quello anche della spartizione del finanziamento pubblico ai partiti.

decreto che conferma il finanziamento delle missioni in cui l'Italia è attualmente impegnata. Vorrei svolgere due osservazioni preliminari. La prima, è che questo finanziamento viene confermato per il primo semestre 2009, anziché con scadenza annuale. In tal modo si consente il costante rapporto con il Parlamento che è stato richiesto in Commissione parlamentare sia al Senato, che alla Camera. L'altra osservazione è che le risorse stanziate dall'Esecutivo risultano di entità consistente, soprattutto rispetto alle misure di contenimento della spesa pubblica che hanno improntato l'ultima manovra finanziaria. È quindi uno sforzo che il Governo ha fatto a riprova della priorità strategica delle missioni internazionali nel quadro della politica estera del nostro Paese.

disposizione ristabilisce su base semestrale uno stanziamento di 45 milioni di euro destinati alla cooperazione allo sviluppo nelle aree di crisi (cioè Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia), al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione civile e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, limitrofi, non trascurando, anzi, impegnandosi anche al sostegno della ricostruzione civile. del nostro Paese si integra così con il sostegno civile alla ricostruzione. Ovviamente, gli effetti benefici sono reciproci e questo viene dimostrato dalla priorità assoluta che il provvedimento assegna

la possibilità per il Ministero degli affari esteri di conferire incarichi temporanei a organismi ed enti specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione purché in possesso di specifiche professionalità, con preferenza, anche in questo caso, per le professionalità locali. Vengono poi potenziate le attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, con un raccordo tra Governo e Parlamento, e con speciale riferimento alla partecipazione italiana, per gli aspetti civili e militari, alle missioni internazionali. Sempre nell'ambito degli interventi a sostegno dei processi di pace, l'articolo 1 del decreto-legge dispone lo stanziamento di circa 10 milioni di euro

nell'ambito di organizzazioni multilaterali, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea. In questo ambito, viene in particolare stanziata una cifra consistente per le missioni NATO di addestramento delle forze armate e di polizia dell'Iraq.

3, reca altresì nei successivi articoli da 4 a 6 le norme relative al personale, nonché quelle in materia penale e contabile. Ciò inquadrato in uno scenario che riguarda gli impegni del nostro Paese in tutte le aree in cui le nostre forze armate sono presenti, ossia nel Medio Oriente, in Afghanistan, nei Balcani ed in Africa. Per quanto riguarda il Medio Oriente, sottolineo che la crisi mediorientale in corso impone un'attenta meditazione della presenza italiana nell'area: il personale militare italiano è presente ad Hebron e a Rafah, ma soprattutto nel Libano meridionale, con la missione UNIFIL, rifinanziata dal decreto. Alla luce dell'evoluzione della situazione nella Striscia di Gaza, è possibile prevedere che possa risultare necessaria una presenza internazionale, anche con la partecipazione dell'Italia per garantire il mantenimento del cessate il fuoco

Ricordo le considerazioni svolte dall'ambasciatore Sequi, rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan, presso la Commissione affari esteri lo scorso 6 novembre in merito alla problematicità delle missioni di pace nella zona. Analoghe preoccupazioni sono state ribadite anche dal Capo di Stato maggiore della difesa, Camporini, nel novembre 2008 e dal Ministro della difesa il 10 dicembre 2008 innanzi alla Commissione difesa. La conferma e anzi l'aumento dell'impegno italiano nella zona costituisce una precisa scelta strategica in linea con i nuovi obiettivi della NATO nell'ottica di dare un segnale di ristabilimento

nell'ambito della missione EULEX per la formazione delle forze di sicurezza kosovare e la tutela di tutte le minoranze presenti. Viene anche confermata la presenza della Guardia di finanza in Libia per il contrasto all'immigrazione clandestina. La Commissione affari esteri ha esaminato il disegno di legge di ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, il quale pone già le premesse per una sempre più stretta relazione bilaterale, soprattutto sul piano della disciplina dei flussi migratori e della politica energetica. Lo abbiamo esaminato la settimana scorsa ed abbiamo sottolineato l'importanza di questo accordo, che non è solo di amicizia, ma è un vero accordo di partenariato fra i due Paesi. Viene aumentato il nostro impegno per la missione in Darfur e contro la pirateria somala e si conferma la partecipazione alla missione in Georgia, deliberata lo scorso anno, seppure permane la problematica relativa al suo effettivo dispiegamento anche in Abkhazia e Ossezia meridionale. Personalmente ritengo condivisibile che l'Italia, nell'anno della presidenza del vertice G8, confermi il proprio impegno nei vari scenari internazionali di crisi,

ma condotta in concorso con le organizzazioni internazionali, segnatamente l'Unione europea e le altre comunità internazionali; è una

Abbiamo votato unanimemente il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e pertanto propongo l'approvazione da parte del Senato di questo provvedimento. *(Applausi

la copertura di 27 missioni, per un periodo di 6 mesi; in ciò si innova rispetto alla situazione precedente, che vedeva l'emanazione di un decreto di copertura annuale. Questo è a mio vero parere un fatto positivo, perché consente una maggiore elasticità da parte del Governo ed anche maggiore possibilità da parte del Parlamento di seguire più da vicino lo sviluppo di tali operazioni. Queste operazioni di pace, che richiedono uno sforzo finanziario non indifferente ed un sacrificio da parte di circa 10.000 cittadini soldati italiani, rischiano

sviluppano - per carità, legittimamente - accesissimi dibattiti su problemi che hanno un loro peso e una loro importanza (della quale non voglio discutere) in ambito nazionale, ma che in ambito internazionale lasciano, se mi consentite, il tempo che trovano. Per converso, quando si parla dell'impegno di 10.000 uomini, ripetuto per un'infinità di anni e per cento missioni in ambito internazionale, si considera il decreto di proroga delle missioni un elemento di *routine* di scarso interesse. A mio parere, questo è un grosso errore di carattere politico una non assunta comprensione di quanto tutti da anni ripetono: la globalizzazione, l'importanza internazionale, le ripercussioni in ogni Nazione di quanto avviene sul piano internazionale. Pertanto, questo mio intervento inizia con l'esortazione di prestare maggiore attenzione a quello che rappresenta, ripeto, il più importante degli interventi internazionali svolti dalla nostra Nazione. Un intervento che determina grandi ritorni non solo da parte dei Paesi occidentali, ma direi da parte dei Paesi di tutto il mondo, in particolare di quelli che vengono interessati dalla nostra azione, con le loro popolazioni ed i loro capi politici o religiosi. Insomma, deve essere fatto a mio parere da parte dalla classe politica italiana uno sforzo di presa di coscienza dell'importanza della partecipazione italiana a queste missioni partecipazione ad operazioni che si protraggono da tempo, nei confronti delle quali dal punto di vista politico l'autorizzazione iniziale ha già visto interessato il Parlamento,

un emendamento, che poi avrò modo di illustrare invitando l'Aula ed il Governo ad accoglierlo, in modo da consentire al Parlamento di dare le opportune indicazioni al Governo nel momento in cui si decide di prolungare le attività ovvero, eventualmente, di iniziarne delle nuove. spunti interessanti di questo decreto sono rappresentati innanzi tutto dal fatto che, mentre in finanziaria è stato assegnato un miliardo di euro per la copertura delle operazioni per l'intero anno,

alle assegnazioni di bilancio per la Difesa ed alle assegnazioni per la Difesa nell'ambito del Ministero dello sviluppo, per cui, in sostanza, anche sul piano internazionale non è giusto affermare che l'Italia spenda decisamente molto meno degli altri Paesi con i quali ci confrontiamo. Se sommiamo tutte queste risorse vediamo che l'Italia fa uno sforzo forse non sufficiente, ma certamente più decoroso di quello che normalmente si crede per la propria Difesa. Debbo dire che ciò da una parte rappresenta un merito dell'attuale Governo e dell'attuale responsabile del Ministero, dall'altra è anche un motivo di soddisfazione

Un secondo aspetto interessante - la novità - è la nostra partecipazione all'operazione antipirateria nell'Oceano indiano. Anche questo è un motivo di soddisfazione per noi,

infine un incremento temporaneo delle forze nell'area balcanica, in particolare per quanto riguarda la Bosnia e in parte il Kosovo. Quindi, sostanzialmente le missioni rimangono quelle di prima. L'entità della partecipazione italiana vede un leggero aumento in funzione di esigenze contingenti qualità delle missioni presenta una leggera evoluzione. Abbiamo iniziato con missioni di carattere esclusivamente militare, condotte soprattutto da forze militari integrate, per la verità, presenza dei Carabinieri, che sono sì militari, ma svolgono soprattutto funzioni di polizia. Oggi ben 12 operazioni sono condotte da forze di polizia, il che in maniera positiva dimostra che vi è una certa evoluzione verso la realizzazione del concetto fondamentale

puramente militare e di sicurezza ad una problematica di sicurezza civile una volta che è stata assicurata la stabilità; a ciò si collega la partecipazione non indifferente di forze di polizia italiane. Un altro indice dell'evoluzione positiva, seppur lenta, è rappresentato dal fatto che cinque missioni sono condotte dalla Guardia di finanza, la quale ovviamente

dall'entità delle risorse che lo Stato dedica alla Difesa e vi è una presenza maggiore di quanto non costi lo strumento militare per l'Italia. La partecipazione alla missione denominata Atalanta è motivo di soddisfazione, come ho detto prima, dal momento che recepisce un invito del Senato al Governo. Viene ancora una volta confermata l'affidabilità che l'Italia con le sue Forze armate e di polizia polizia ha in ambito internazionale in situazioni difficili, ad alto rischio, spesso drammatiche sia per le popolazioni che per i nostri operatori.

una forza di carattere politico e professionale, una forza umanitaria, una forza di pace e stabilizzazione contro le minacce terroristiche (di cui tutti parlano) e sovvertitrici della democrazia.

andare la nostra stima per la loro capacità professionale, lo spirito di sacrificio ed il coraggio, nonché la nostra gratitudine per l'azione di prevenzione e di tutela dai pericoli e dalle minacce, non solo a favore delle popolazioni soccorse, ma, in una visione

non può che compiersi secondo il dettato costituzionale e secondo le direttive dell'ONU, cioè coniugando il tema della sicurezza internazionale con quello dello sviluppo e dell'autonomia dei territori oggetto del nostro impegno. In particolare, voglio fare riferimento alla situazione afgana, nella quale da sempre sosteniamo che il processo di pace non può che venire da un'azione congiunta che sia anche militare ma non solo militare. caso è altresì necessaria una decisa iniziativa politica per affrontare le grandi priorità che rendono insostenibili le condizioni di vita della popolazione locale. cento di questa vive sotto la soglia di povertà e i dati ufficiali ci dicono che il 70 per cento non ha un lavoro legale e il 60 per cento non dispone di energia elettrica. cento della popolazione adulta non va oltre l'istruzione elementare e il tasso di analfabetismo femminile è dell'85 per cento. È poi la popolazione civile a soffrire di più per gli insulti delle armi. Solo per citare un caso, ricordo che gli attacchi aerei della missione *Enduring* *Freedom* sono stati la causa principale, ancorché involontaria, di morti civili e danni alle proprietà. Si tratta di una situazione che ha diffuso la percezione che si sia indifferenti alle vittime civili e che non si facciano abbastanza sforzi per proteggere i cittadini e le loro proprietà durante le incursioni. Oltre sette anni dopo la fine del regime dei talebani e l'inizio dell'intervento internazionale, le notizie che giungono da quel Paese non lasciano molto spazio all'ottimismo. Tuttavia, in questi sette anni sono stati raggiunti risultati importanti, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione delle istituzioni, la ripresa del settore sanitario e di quello scolastico, lo sviluppo di quello dell'informazione. Molte, però, sono ancora le difficoltà, a partire dalla sicurezza in continuo deterioramento, nonostante la presenza di truppe internazionali. C'è la lentezza della ricostruzione dello sviluppo economico, ancora non in grado di migliorare lo stato di diffusa povertà della popolazione. C'è poi la perdurante piaga della coltivazione e del traffico di oppio arrivati, in questi anni, a livelli mai raggiunti in passato. Coltivazione e traffico di droga andrebbero finalmente contrastati, essendo il bacino afgano il più grande del mondo. Nei nuovi livelli di governo delle istituzioni appare resistere inoltre, a giudizio degli esperti, la cultura dell'impunità:

laddove le elezioni politiche, hanno visto una partecipazione del 50 per cento. Quel Paese manifesta il bisogno di una strategia di lungo periodo, che affronti i nodi trascurati di una *governance* inefficace e priva di visione, che adotti tutte le misure utili a punire i responsabili dei fenomeni di corruzione, a partire da quelli del narcotraffico. Al tempo stesso, è urgente favorire l'emersione di una società civile e politica che possa consentire il ricambio; si tratta di una società civile e politica che ora appare schiacciata da dinamiche economiche e di potere fortemente legate alla guerra. Tra l'altro, secondo una serie di recenti studi, i principali donatori della comunità internazionale portano la responsabilità dei fallimenti attuali sulla ricostruzione. Questo sia perché manca una visione coordinata degli interventi, sia perché solo il 40 per cento delle risorse rimane in Afghanistan, mentre il 60 torna ai Paesi donatori attraverso le loro ONG e le agenzie private per lo sviluppo. Per quanto riguarda l'impegno fin qui sostenuto dall'Italia in Afghanistan, questo è stato principalmente dettato dalle scelte di solidarietà transatlantica, piuttosto che da un sentimento di reale interesse nazionale. Sin qui l'Italia, in linea con quanto facevano gli Stati Uniti, ha devoluto il 90 per cento dei propri finanziamenti all'Afghanistan alla sfera militare, con ciò lasciando molto poco all'impegno della cooperazione internazionale. Voglio dare credito a quanto il sottosegretario Scotti ci ha detto nell'ultima audizione in Commissione diritti umani. Scotti ha sostenuto che l'impegno del Governo italiano a favore dei diritti umani è una componente trasversale della nostra azione internazionale; il Parlamento ed il Governo dichiarano di condividere, infatti, una politica di promozione dei diritti umani fondamentali della persona, tanto che esiste - a detta di Scotti - una sensibilità sempre più diffusa secondo cui la democrazia e i diritti umani sono componenti essenziali della nostra azione nel mondo, al punto da tracciare una via italiana all'impegno in politica estera. Per questi motivi, cosi velocemente e sinteticamente enunciati, sono rimasta negativamente colpita dal fatto che la maggioranza e il Governo abbiano bocciato in Commissione tutti i nostri emendamenti, che avevano principalmente il fine di integrare, peraltro assai modestamente, ma almeno simbolicamente, le risorse sul fronte degli aiuti alla popolazione civile afgana; quella popolazione verso la quale dovremmo rivolgere il massimo della nostra attenzione, anche perché essa, troppe volte, è risultata vittima innocente degli insulti delle armi.

Abbiamo presentato oggi una mozione su questi temi: allora perché in questo atto non c'è neanche un euro per iniziare un'opera di prevenzione vera delle mutilazioni dalle mine e dalle *cluster bomb*? Perché oggi in quest'atto non c'è neanche un euro per la restituzione ai civili di un territorio sanato? Credo che se vorremo essere coerenti e credibili con il mondo, oltre che con la nostra coscienza - bene prezioso e sempre più raro, ma irrinunciabile - dovremo pretendere un impegno diverso e maggiormente caratterizzato sul fronte della politica e della cooperazione internazionale. il dibattito che ha accompagnato fin qui l'esame del provvedimento alla nostra attenzione ha messo in evidenza, tra l'altro, l'opportunità di stabilire un percorso parlamentare tale da consentire un approfondimento sulle linee politiche fondamentali in materia di partecipazione italiana alle missioni internazionali. Lo ricordava il relatore, senatore Ramponi, e a questo proposito voglio citare l'intervento svolto davanti alle Commissioni 3ª e 4ª riunite dal sottosegretario Mantica, Si tratta quindi, a ben vedere, di un'opportunità da perseguire con convinzione e decisione, anche per evitare il rischio, sempre presente, che l'approvazione di così importanti provvedimenti si trasformi in un semplice adempimento burocratico. D'altra parte, così non è né dovrà essere in futuro. Mentre discutiamo, infatti, circa 8.500 uomini e donne sono impegnati, anche a rischio della propria vita, nei diversi scacchieri internazionali, caratterizzati da condizioni sempre critiche e particolarmente difficili. ufficiali e militari di truppa che in questo momento sono lì a rappresentare con coraggio e dignità il nostro Paese. Nel riaffermare con forza ai nostri connazionali impegnati nei diversi scenari di crisi tutta la nostra stima e tutto il nostro sostegno, non possiamo però evitare di sottolineare il carattere tutto politico sotteso all'assorbimento di questi gravosi impegni da parte del nostro Paese. Garantire il contributo dell'Italia alla comunità internazionale per la stabilizzazione e la ricostruzione di aree di crisi non può essere affidato, infatti, unicamente alla presenza militare, al cosiddetto impegno operativo. Si deve agire contemporaneamente con la messa in campo di strumenti, risorse e politiche che sappiano aiutare le comunità interessate a costruire le migliori condizioni per la realizzazione di una transizione sicura e stabile. Così penso possiamo davvero proiettare nello scenario internazionale il ruolo del nostro Paese sul fronte di un multilateralismo concreto ed efficace. Se questo può risultare un asse condiviso di ragionamento e di conseguente azione di politica internazionale, appare del tutto evidente che il Parlamento non può limitarsi ‑ credo ad affrontare così delicate questioni in una discussione che si limiti ad approvare un decreto‑legge di rifinanziamento delle missioni. Vi è bisogno, invece, di un confronto di merito più profondo, che interessi in modo compiuto tutti gli aspetti politici riguardanti il nostro impegno internazionale, anche al fine di promuovere una solida coesione su temi così delicati, che riguardano l'interesse generale del nostro Paese nel contesto internazionale. Gli argomenti di approfondimento e di confronto politico di merito, certo, non mancano: penso, ad esempio, alle questioni più delicate, che afferiscono al nostro impegno, quali l'Afghanistan o lo scacchiere mediorientale. È necessario, quindi, che la procedura sia rivista, individuando altre modalità, non limitando il confronto parlamentare all'esame delle singole, specifiche autorizzazioni di spesa. Ed è proprio su questo argomento che vorrei, infine, svolgere alcune considerazioni, relativamente alla congruità delle risorse messe a disposizione dal provvedimento. In primo luogo, si osserva che il provvedimento al nostro esame ripropone ‑ come già sperimentato nella XIV legislatura ‑ un rifinanziamento per un solo semestre, da rinnovare a metà dell'anno per un periodo della stessa durata. Questo afferma il Governo per dare maggiore flessibilità all'impiego delle risorse. Nel merito delle cifre e dell'entità del finanziamento, così com'è stato modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, la maggioranza sostiene di avere dato risposta alla necessità di destinare appropriate risorse finanziarie alle nostre missioni internazionali, presentando il quadro complessivo dei fondi destinati incrementato di circa il 30 per cento rispetto al precedente finanziamento. In realtà, come detto, l'intervento finanziario riguarda il primo semestre del 2009 e introduce tra l'altro nuovi impegni, nuove missioni, rispetto all'anno precedente. Si potrà parlare, quindi, di un incremento di risorse soltanto a conclusione del periodo annuale, tenuto conto che al momento risulta messo a disposizione circa il 70 per cento dei fondi previsti per il 2009 dalla finanziaria approvata a suo tempo dall'allora Governo di centrosinistra. Si pone perciò alla nostra attenzione il necessario reperimento di ulteriori e adeguati fondi per la partecipazione italiana alle stesse operazioni per il secondo semestre dell'anno. Anche su tale questione, che può apparire di semplice natura tecnica, credo torni alla ribalta il tema di un esame più preciso e approfondito da parte del Parlamento dei provvedimenti concernenti la nostra partecipazione alle missioni internazionali. Auspico, signor Presidente, che i prossimi mesi possano essere ben utilizzati proprio a questo scopo.

o del Gruppo. Il disegno di legge n. 1334, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, costituisce, nel riproporsi periodicamente, ogni semestre, un atto di quelli che potremmo indicare quasi come dovuti, al pari della legge finanziaria o delle leggi di bilancio, nel nostro programma legislativo. È prassi invalsa, infatti, che ogni sei mesi, data la necessità di assicurare la continuità delle missioni internazionali, si preveda il rifinanziamento delle stesse e, sempre nella medesima *ratio*, dato il mutare degli scenari internazionali, si disponga parimenti l'integrazione degli impegni all'estero, ovvero la riduzione e la rimodulazione degli stessi.

mio e del mio Gruppo alla discussione in Commissione esteri e a quella odierna in Aula non è volto a fare opposizione ma esclusivamente al miglioramento del disegno di legge di conversione. In tal senso abbiamo presentato due ordini del giorno, che servono a mettere in luce possibili problematiche sulle quali un impegno del Governo potrebbe risultare fondamentale. Il primo attiene alla disposizione che autorizza il Ministero degli affari ad affidare consulenze esterne, nonché alla relazione semestrale che lo stesso Ministero è tenuto a presentare alle Camere; il secondo riguarda la copertura finanziaria del provvedimento. su questo tema, signor Presidente, mi riservo di intervenire, insieme al collega Caforio, nella sede specifica dell'illustrazione degli ordini del giorno. Per quanto attiene al disegno di legge, invece, vorrei soffermarmi sugli aspetti di maggiore rilevanza per il Ministero degli affari esteri, specificamente gli articoli 01, 1 e 2. L'articolo 01, 2. L'articolo 01, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, introduce nella norma un capitolo concernente gli interventi di cooperazione allo sviluppo e costituisce, a mio avviso, un importante contributo parlamentare alla disposizione governativa, dimostrando in tal modo che il Governo dovrebbe avvalersi maggiormente del contributo delle

per giocare un ruolo determinante anche in quelle situazioni post conflitto, nelle quali le infrastrutture di base, i servizi pubblici minimi e la funzionalità di un sistema complessivo, sia economico sia politico, sono stati indeboliti dal protrarsi delle ostilità. In particolare, nel disegno di legge n. 1334 si stabiliscono interventi in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, specifici per la ricostruzione e l'assistenza ai rifugiati. Si assegna per tali interventi un fondo di 45 milioni di euro che va a modificare quanto disposto nella legge finanziaria per il 2009. Vorrei ricordare che, proprio su tale aspetto, a dicembre 2008 la discussione relativa alla manovra finanziaria mi aveva visto condurre una decisa opposizione in Commissione affari Infatti, quello che si disponeva in finanziaria, alla Tabella C allegata alla legge, era una riduzione progressiva e costante, a partire dal 2009 e fino al 2011, dell'impegno economico dell'Italia. Per essere precisi, si prevedeva una riduzione pari a 500 milioni di euro per il 2008 e di ulteriori 100 milioni nel 2011. Non possiamo, quindi, che accogliere positivamente questa parziale inversione di rotta che riduce il taglio ignominioso stabilito a dicembre. Rifinanziare le missioni di cooperazione allo sviluppo è importante, infatti, non soltanto per non perdere di credibilità nei confronti di quelle popolazioni che fanno affidamento sul contributo italiano, nonché nei confronti dei partner stranieri con i quali cooperiamo nei teatri di Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, ma è fondamentale anche per sviluppare appieno la nostra politica estera. Le missioni all'estero, per come si configurano attualmente, coniugano sempre di più l'aspetto militare della difesa, ossia il *peace keeping*, a quello umanitario, cioè il *peace building*. È chiaro

di raggiungere risultati concreti sono basate non più sulla mera forza di interposizione ma sullo sviluppo di relazioni con le popolazioni autoctone, sull'instaurazione di un clima di fiducia, sul ripristino delle strutture essenziali e sulla legittimazione dei Governi locali. Sono basate, insomma, su di un'attività che riesce gradualmente a restituire l'autonomia di gestione al Paese in cui operiamo per poter sganciare la presenza straniera sul territorio e passare la consegna ad istituzioni interne forti e ad una società civile pacificata. Per tali motivi riconoscere l'importanza della cooperazione allo sviluppo ed incentivare, come si fa al comma 2 dell'articolo 01, l'utilizzo delle risorse locali sia umane che materiali costituiscono un passo importante. Il panorama delle attività con le quali l'Italia contribuisce al mantenimento della pace è arricchito poi dall'articolo 1, ove si stabiliscono gli interventi per le esigenze di prima necessità, come il ripristino dei servizi essenziali, della popolazione locale di Libano, Afghanistan e Balcani. Considerando che tali interventi possono essere stabiliti dai comandanti dei contingenti militari impegnati nei suddetti teatri, si deve rilevare che la disposizione permette elasticità e prontezza di azione, rispettando il principio della vicinanza dei centri decisionali alle situazioni da gestire. Passando successivamente all'analisi dell'articolo 2, concernente gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si deve innanzitutto notare come lo spirito multilaterale della politica estera italiana sia rafforzato e come si vadano a privilegiare nuovamente strumenti alternativi a quelli militari per la creazione di uno spazio di pace e sicurezza: nello specifico, i fondi fiduciari NATO, la diplomazia preventiva OCSE e la partecipazione di funzionari alle missioni PESD, la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea. per i quali si assegnano due milioni e mezzo di euro, sono utilizzati per sostenere le istituzioni dei Paesi partner indebolite dalle guerre, mentre il ruolo italiano in ambito OCSE si svolge su più fronti, dal controllo sul rispetto degli accordi di pace e sullo svolgimento delle consultazioni elettorali (per le quali l'Italia impegna 40 esperti) alla lotta alla criminalità internazionale e alla corruzione. A conclusione di quanto detto sinora, il giudizio sulle missioni italiane, di carattere se vogliamo civile, non può che essere positivo ed anzi, si auspica che tale aspetto della nostra politica estera, il quale coniuga la solidarietà globale con la presenza sul territorio, possa essere sempre più di primo piano. Tale sfera della politica estera appare imprescindibile altresì come strumento per rafforzare la posizione italiana nei consessi internazionali, Europa, NATO, ONU, OCSE, e per poter offrire, in caso di recrudescenza delle conflittualità, non soltanto contingenti militari ma pieni rapporti di collaborazione politica con i governi interessati e profonda conoscenza delle condizioni dei civili.

Senza entrare nello specifico delle singole missioni, mi soffermo nel sottolineare solo che il comma 25 dà attuazione al Trattato di amicizia con la Libia, che è stato da parte dell'Italia dei Valori fortemente contestato, in quanto manchevole delle giuste clausole di salvaguardia dei diritti umani. Lo rimarchiamo ancora oggi, perché è un interesse di parte, per quanto riguarda l'Italia dei Valori, e lo vogliamo dire forte Voglio quindi rilevare la sensazione generale sorta dalla lettura dei 33 commi: mi sembra che il quadro sia caratterizzato da un'eccessiva varietà e diffusione delle missioni, e manchi spesso di consistenza delle stesse. Si legge, ad esempio che nella missione ad Haiti, la MINUSTAH, sono impegnate cinque unità della Guardia di finanza. nel senso che, per conseguire risultati effettivi, si sarebbe forse dovuto procedere a una razionalizzazione delle forze militari all'estero e a una riallocazione degli impegni laddove questi sono più richiesti. Questo farà parte dell'ordine del giorno Per concludere, cari colleghi, vorrei sottolineare ancora una volta come all'Italia dei Valori stia a cuore il dovere di proseguire negli accordi multilaterali presi, e di assicurare la massima sicurezza per i nostri militari impegnati all'estero. Pertanto, dimostriamo con spirito di collaborazione il nostro impegno per il rifinanziamento delle missioni. Vorrei, e concludo con questo monito, che si prestasse un'attenzione particolare perché l'efficacia delle missioni risiede proprio nella possibilità di mantenere una continuità ed un livello di prestazioni alto nel tempo, mentre una gestione improvvida delle finanze pubbliche, senza programmaticità

muovo da quelle stesse preoccupazioni che il relatore, senatore Ramponi, illustrava nel corso del suo intervento, e cioè che un atto così importante per il nostro Paese, come sono le missioni internazionali e le decisioni che le riguardano, avvenga senza un reale approfondimento delle condizioni politiche nelle quali queste missioni si svolgono, senza un bilancio e una valutazione delle diverse situazioni e dei diversi scenari nei quali i soldati italiani sono impegnati, in sostanza senza che il Parlamento svolga il ruolo che gli è proprio, di esercitare una funzione di indirizzo. Vorrei sottolineare che questa preoccupazione è particolarmente rilevante, intanto perché siamo in una fase di profondo mutamento degli scenari e delle situazioni; in una fase nella quale è aperta, in tutti i Paesi che insieme a noi hanno la responsabilità di queste missioni, una discussione politica sulle scelte che devono essere compiute. In secondo luogo

La Russa, esprimeva profonda preoccupazione ed allarme sulle condizioni nelle quali i nostri soldati e le nostre forze sono impegnate. Mi pare che questo sia un problema essenziale e credo che attraverso l'odierna discussione dobbiamo contribuire a tracciare questo quadro e questo indirizzo. Mi soffermerò, in particolare, sulla missione italiana in Afghanistan non perché sia l'unica ma perché, osservando questa missione e i problemi che ha di fronte,

la situazione in Afghanistan è rischiosa. Leggo proprio adesso su un'agenzia che questa mattina a Kabul, in coincidenza con la visita

territorio afgano, ad abbandonare l'Afghanistan dichiarando che non esistono più le condizioni per garantire i livelli di sicurezza necessari.

le forze e le persone lì impegnate e, più in generale, il destino di questa missione e dell'intervento della comunità internazionale per riaffermare condizioni di stabilità e sicurezza in quella regione.

il contesto nel quale si svolge la missione italiana; è un contesto nel quale i fenomeni di corruzione non diminuiscono, nel quale la base politico-sociale del governo Karzai, che dovrebbe garantire una crescita della stabilità politica, non si allargava, nel quale i dati ci dicono che la produzione e il traffico di stupefacenti, la coltivazione del papavero e dell'oppio e la produzione di eroina continuano a crescere in modo inarrestabile. È una situazione nella quale ‑ voglio ricordarlo ‑ nel corso di questo anno sono stati uccisi oltre 2.100 civili e di questi più di 800 sono stati uccisi non dai talebani, ma in operazioni condotte o dall'esercito afgano o direttamente dalle forze militari internazionali.

conquista dei cuori e delle menti, cioè la conquista di quelle condizioni politiche che potevano permettere un successo dell'iniziativa), appare sempre più in difficoltà.

tra chi pensa che in Afghanistan sia possibile semplicemente una soluzione militare (e, di conseguenza, orienta in questo modo i comportamenti delle forze ivi presenti) e chi ritiene che l'azione militare debba avere un ruolo di garanzia delle condizioni di sicurezza che permettono di sicurezza che permettono alla politica di svilupparsi. Ma questo è un punto sul quale il nostro Paese può esercitare un ruolo. Tutti noi dobbiamo avere il senso delle proporzioni, di quello che l'Italia è e può fare, ma in una situazione di trasformazione, nella quale nella nuova amministrazione americana è nata una riflessione sulle strategie da seguire, il nostro Paese, nel quadro delle relazioni internazionali e degli impegni internazionali che assume, può esercitare un ruolo, può spingere e premere per una politica, e lo può fare in modo più efficace costruendo, se costruendo, se riesce, un collegamento e una omogeneità tra i diversi Paesi europei che in quegli scenari sono impegnati. convinzione il rinnovo del mandato e del finanziamento alle nostre missioni, però pensiamo che oggi ci sia un'azione del Governo radicalmente insufficiente dal punto di vista

sappia e abbia coscienza di come sia importante non essere sconfitti in Afghanistan e di come invece questa sia una possibilità che oggi concretamente si presenta. Infine, voglio ricordare - perché

In Pakistan, come abbiamo letto in questi giorni, è stato raggiunto un accordo con i talebani ed il punto di compromesso è stato l'applicazione della *sharia*

in una possibile politica di stabilizzazione della situazione afgana. Questi pare a noi siano i problemi

di un Parlamento che sia in grado di dare una valutazione politica e di esprimere un indirizzo e di un Governo che permetta all'Italia...

come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduta, il provvedimento in discussione ha ad oggetto unicamente il rifinanziamento delle missioni in corso e non si presta al dibattito approfondito che il Parlamento dovrebbe invece svolgere sugli aspetti politici inerenti alle missioni internazionali e in particolare, come ha sottolineato il senatore Marcenaro, ai punti più evidenti di crisi come l'Afghanistan, ma potremmo anche dire al mantenimento della pace in Libano.

rafforzare il nostro contingente in Afghanistan, forse di cambiare le regole di ingaggio, forse di implementare anche le missioni umanitarie e civili; leggiamo, in una dichiarazione rilasciata proprio ieri dal ministro La Russa, che forse dovrà sottoporre un ulteriore provvedimento a questo Parlamento. Allora chiediamoci perché non siamo in grado oggi di fare quello che il senatore Ramponi chiedeva, cioè calamitare l'attenzione politica e di questo Parlamento su quello che stiamo facendo oggi.

sono state avanzate almeno tre proposte per modificare l'approccio, il tipo, il senso politico di questo nostro lavoro di rifinanziamento con decreti. Alcuni di noi hanno proposto di individuare un nuovo metodo, come quello di una legge quadro periodica, per l'approvazione degli atti legislativi di rifinanziamento, in modo che il Parlamento possa incidere più efficacemente.

ci soddisfa solo in parte. Sottosegretario Cossiga, vorrei riflettere sul motivo della sua freddezza su questo nodo, quando lei rispose in Commissione

il metodo di valutazione politica del coinvolgimento del Parlamento sul nodo delle missioni, così come avviene peraltro nel Parlamento americano. Questa separatezza burocratica non ha più ragion d'essere.

la partecipazione alle missioni internazionali colloca il nostro Paese tra i maggiori contributori di forze che operano nei teatri operativi di quattro continenti diversi. Questa partecipazione è ed è stata sempre subordinata a criteri molto qualificanti: la multilateralità dell'intervento, la legittimazione del mandato, il rispetto assoluto dei costumi delle popolazioni. Ma, soprattutto, l'impegno italiano è stato costantemente caratterizzato da una specificità: la capacità di collegare l'attività militare con l'azione umanitaria, con gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture e del tessuto sociale e con il sostegno alle istituzioni democratiche. Oggi il decreto all'esame ci ripropone quindi l'approvazione dell'impegno finanziario di tali attività all'estero. sarebbe stato più utile per il rilievo della materia e più consono all'alta funzione di questa Assemblea discutere non solamente l'aspetto finanziario delle missioni, piuttosto esprimere valutazioni in merito alla loro rispondenza; verificare se sono stati compiuti progressi reali verso le condizioni che possono segnare la fine dell'impegno operativo; elaborare modifiche alla strategia delle missioni per renderle, quando necessario, più adeguate alla situazione politica e militare dell'area interessata. In sostanza, sarebbe opportuna l'attribuzione al Parlamento della responsabilità della periodica definizione delle linee politiche ed evolutive dell'impegno dell'Italia nelle missioni all'estero. Mi auguro che questa esigenza, che da più parti è stata sollecitata, venga accolta. Tornando all'esame dell'aspetto finanziario, registro il fatto che le risorse stanziate nel decreto coprano anche le esigenze della preparazione delle unità. Non posso, peraltro, non rilevare come quelle risorse corrispondono buona parte del totale previsto per tutto il 2009; è quindi un impegno obbligato per il Governo adeguare il fondo annuale, per assicurare, anche nel secondo semestre, la disponibilità delle stesse risorse previste per i primi sei mesi. Lo spettro delle missioni che il decreto propone di rifinanziare è molto ampio e differenziato. Peraltro, in termini di consistenza e soprattutto di complessità, il teatro di intervento più rilevante è senza dubbio quello dell'Afghanistan. Ed è proprio sul caso dell'Afghanistan che vorrei soffermarmi brevemente. In quel Paese, il quadro di situazione è caratterizzato, più che nel passato, da un'accentuata complessità. I risultati conseguiti negli ultimi sette anni hanno riavviato un processo di pace nella Nazione, dopo tre decenni di guerra, ma tali risultati non appaiono ancora definitivi e soprattutto non appaiono consolidati. Il processo di stabilizzazione è fortemente minacciato dall'insorgenza, dalla criminalità, dalle spinte centrifughe dei poteri regionali, dalle influenze delle Nazioni dell'area, confinanti o no. L'Italia è chiamata a continuare la sua opera, insieme alle altre 40 Nazioni contributrici di forze. Ma l'azione militare, essenziale per rafforzare l'autorità del Governo afgano e per sostenere le forze militari e di polizia, non può, né potrà, essere risolutiva. Occorrerà affiancare all'intervento militare, ancor di più di quanto fatto finora, una forte azione per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni. In Afghanistan, più che negli altri teatri, non è pensabile ottenere i risultati a cui tende la comunità internazionale se non si riesce ad acquisire il consenso della popolazione. In questo quadro, credo che le capacità e l'approccio evidenziati dall'Italia in tutte le missioni di supporto alla pace possano costituire un riferimento importante per condurre a compimento una missione difficile e complessa come quella nel Paese asiatico; e credo che l'Italia, in virtù del forte impegno sempre profuso in quel Paese, possa e debba svolgere una funzione promotrice per una nuova e più incisiva strategia. incisiva strategia. Tornando all'insieme delle missioni in esame, ho, infine, il convincimento che una grande riconoscenza debba essere espressa da questo Parlamento e da tutta la Nazione nei confronti dei quasi 9.000 militari e dei civili che, correndo continuamente gravi rischi per la propria incolumità, continueranno, nell'anno in corso, a rappresentare l'impegno dell'Italia per la promozione della pace e per la legalità internazionale. Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per ribadire, a nome di tutto il Gruppo Italia dei Valori, che riconosciamo pienamente l'importanza della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali in generale. Siamo infatti convinti che non si possa prescindere da esse se si vuole perseguire una politica concreta di cooperazione in materia di affari esteri, difesa e, più in generale, di sicurezza per il nostro Paese. Come tutti i colleghi sanno, questo fine è uno dei più importanti tra quelli che ci si pone anche a livello comunitario ma, nelle more di un maggiore, e da sempre da noi auspicato, rafforzamento della politica estera e di difesa a livello europeo, capiamo bene che il prestigio dell'Italia a livello internazionale dipende dalla sua adesione ai Trattati istitutivi di organismi internazionali o sopranazionali di cui è membro. Per questi motivi, colleghi, sarebbe molto difficile sostenere tesi o comunque argomentare contro l'utilità di dette missioni. Siamo infatti persuasi della necessità e utilità delle missioni in cui sono impegnati attualmente i nostri militari. Così come siamo persuasi del fatto che che il nostro impegno nelle Aule parlamentari debba essere sempre volto a rendere il loro ruolo il più efficace possibile e le loro missioni le più risolutive, garantendo al massimo livello la sicurezza di tutti i nostri operatori. Ciò non toglie, però, colleghi, che il nostro Gruppo voglia dire la sua sulla modalità con la quale queste missioni vengono decise e sistematicamente proposte. Cogliamo, infatti, con favore il fatto che i colleghi della Camera abbiano approvato una modifica all'iniziale formulazione del decreto, prevedente appunto il finanziamento di una politica quale quella della cooperazione al fine nobile dello sviluppo, importantissima per il mantenimento della pace e più in generale del miglioramento delle condizioni di vita dei civili che hanno avuto la sfortuna di nascere e vivere in scenari di guerra e di particolare disagio. L'auspicio del nostro Gruppo è che si approvi un ulteriore aumento di fondi da destinare alla cooperazione allo sviluppo, per consentire che l'intervento militare possa svolgersi in condizioni più tranquille e più sicure soprattutto in quelle parti del mondo dove l'aiuto sarebbe più necessario. Apprezziamo, quindi, che la Camera abbia portato all'introduzione di tale voce di spesa, ma riteniamo che la cifra stabilita non sia ancora sufficiente ai fini dell'attività. Siamo poi piuttosto preoccupati - credetemi, colleghi, lo dico senza alcuna falsa retorica - per diverse questioni che risultano, ad oggi, poco chiare. In particolare, all'Italia dei Valori farebbe piacere sapere qual è la linea che il Governo intende seguire soprattutto in relazione alle importanti missioni in Medio Oriente a cui l'Italia partecipa lo avrete capito - al delicatissimo impegno in Afghanistan: non si può non essere preoccupati in merito ad una missione in cui l'Italia impegna il maggior numero di soldati), missioni al cui riguardo, lo ricorderete, si è discusso nei mesi scorsi allorquando parve necessaria una rimodulazione dei cosiddetti *caveat*. Ancora, colleghi, ricorderete le forti preoccupazioni manifestate da più parti in occasione della discussione sull'ultimo decreto di rifinanziamento di dette missioni in seno a questa Assemblea, nonché dai colleghi in Commissione difesa circa l'impiego dei nostri Tornado. Preoccupazione, converrete con me, fondata e avvalorata adesso anche dal testo di questo decreto. La situazione in Afghanistan, come tutti sappiamo, è sempre più delicata e anche dal confine pachistano le notizie più attuali non sono confortanti. Basti pensare alla recente notizia circa la richiesta, molto probabilmente a breve accordata, di riconoscere come legge dello Stato addirittura la *sharia*. In questo quadro l'Italia dei Valori, non tirandosi indietro di fronte alle responsabilità riguardanti l'importantissima politica estera e di difesa da perseguire, richiede al Governo, approfittando del decreto per il rifinanziamento delle missioni internazionali, di spendere una parola chiara e definitiva su questo argomento. Un'altra forte preoccupazione per l'Italia dei Valori è rappresentata dalla scarsezza di copertura finanziaria a cui andiamo incontro per l'anno 2009. Come molti in quest'Aula sanno, il capitolo di spesa che riguarda la copertura economica delle missioni del nostro Paese presso Stati esteri è pari a un miliardo per anno. Ebbene, colleghi, il decreto che ci accingiamo a convertire oggi prevede una spesa, solo per il primo semestre, di più di 800 milioni di euro. Va da sé che, non prevedendosi all'orizzonte grandi svolte politiche internazionali tali da poter giustificare una riduzione dei costi per le nostre missioni, sino a stare dentro - passatemi il termine - alla somma residua prevista a bilancio per l'anno in corso, allora converrete con me che qualche dubbio sorge. Per questo, colleghi, pur certo che il Governo saprà trovare giustificazione ed adeguata copertura all'operato dei nostri ragazzi in giro per il mondo, mi chiedo e vi chiedo: non avremo quindi elevato di quasi il doppio la spesa necessaria al mantenimento in vita di dette missioni? non volendo condannare tale effetto, non potremmo qui in quest'Aula, con l'aiuto del Governo che è il proponente di questi disegni di legge, approfittare dell'occasione dataci per discutere seriamente sulle modalità, sui criteri che spingono il nostro Stato a decidere di incrementare così tanto i fondi che si destineranno a tali scopi? il mio non è un processo alle intenzioni del Governo, anzi; c'è solo la mera preoccupazione, fondata, che facendo i "conti della serva" non ci staremo e quindi, per garantire l'incolumità dei nostri ragazzi, dovremo necessariamente allungare la coperta. Però la coperta - non lo dico io, lo raccomandano tutti da sempre - non è bello allungarla per decreto; sarebbe molto meglio una seria e pacata discussione, non di una mattinata come oggi, circa il metodo da voler seguire per il futuro. Per questi motivi, colleghi, colgo l'occasione per annunciare che il Gruppo Italia dei Valori ha inteso presentare solo due ordini del giorno che con il collega senatore Pedica più innanzi vorrei illustrare e su cui spero possa giungere il parere favorevole del Governo, con i quali, appunto, chiediamo che ci sia più trasparenza sui costi delle missioni, le loro finalità, i risultati raggiunti e l'impiego - che, appunto, vorremmo davvero trasparente - di consulenze esterne, come quelle previste dal decreto che ci accingiamo a convertire. Concludo, colleghi, sottolineando il più totale disinteresse dell'Italia dei Valori a mettere in atto pratiche ostruzionistiche di alcun tipo e manifestando la più ampia disponibilità ad affrontare la tematica in questione nelle sedi proprie, quali ad esempio le Commissioni competenti, al fine di poter meglio valutare il da farsi in un campo delicatissimo qual è quello di che trattasi, alla luce delle importanti sfide internazionali a cui il nostro Paese di continuo è chiamato a rispondere.

avviene alla scarsa presenza dei senatori della maggioranza e sicuramente in assenza dei presidenti delle Commissioni affari esteri e difesa. Stiamo discutendo probabilmente dell'unica chiara politica politica internazionale del Governo Berlusconi. Infatti, se dovessimo riassumere per sommi capi quali sono le caratteristiche del nostro impegno in quello che il ministro Frattini all'inizio della legislatura chiamò «multilateralismo efficace», ci sarebbe una grossa difficoltà a non includere, nel novanta per cento degli esempi di questo multilateralismo efficace, la nostra presenza e la partecipazione alle missioni internazionali decretate da organismi regionali o internazionali.

fino ad ora manifestata dai banchi della maggioranza. Il voto che ci accingiamo ad esprimere credo che vada preso in considerazione sotto almeno due punti di vista, il primo relativamente al sostegno che noi dobbiamo mantenere, se possibile anche rafforzare, nella qualità del modo con cui articoliamo gli argomenti a favore della presenza dei nostri contingenti in missioni internazionali; l'altro - ripeto - inquadrandolo all'interno di una politica estera del nostro Paese. Se non fosse stato per il recupero di 45 milioni di euro da dedicare alla cooperazione internazionale, la delegazione radicale del Gruppo del Partito si sarebbe astenuta, non perché contraria alla partecipazione degli italiani nelle missioni internazionali, ma proprio per tutti gli argomenti elencati negli interventi dei senatori del Gruppo del Partito Democratico che mi hanno preceduto.

durante la discussione presso le Commissioni riunite, è stato più volte sottolineato che la parcellizzazione della nostra presenza all'interno di varie missioni non necessariamente può essere considerata una vera e propria scelta politica. Purtroppo si tratta,

detto. Considerato che si tratta di razionalizzare e, proprio per la qualità della partecipazione italiana, di concentrarsi laddove i teatri sono più complessi, probabilmente fare piccole economie e quindi prestare maggiore attenzione alla alla distribuzione dei nostri militari potrebbe andare ad ulteriore sostegno di quanto viene fatto in giro per il mondo. Il problema, però, come è stato sottolineato più volte, da ultimo dal senatore e generale Del Vecchio, è che non si può pensare di portare la pace esclusivamente attraverso la presenza militare. In particolare, il teatro afgano è quello che presenta più problemi. Proprio per cercare di affrontare alcuni di essi

dopo mesi e mesi di grande lavoro di *intelligence*, sono riusciti a sequestrare un quantitativo che sarebbe stato destinato ai mercati della droga in Europa. Ebbene, 700 militari, nell'economia della presenza di un contingente nazionale, sono una quota che viene distolta dalla ricerca dell'affermazione di un minimo di stabilità per portare avanti iniziative di tipo economico, sociale e culturale, quindi pienamente politico destinandola alla cosiddetta guerra alla droga.

con un atto di coraggio e di attenzione alla necessità di fornire analgesici ai Paesi poveri ed in via di sviluppo, essere legalizzata, consentendo la conversione del papavero in morfina e codeina e in una quantità di altre medicine legali (tra l'altro senza neanche brevetto) che potrebbero essere distribuite, attraverso un apposito fondo delle Nazioni Unite, in Africa, in Asia centrale o anche nel Sud delle Americhe, per combattere malattie le più varie semplice, banale operazione alla cura del cancro, che sappiamo essere ormai diventato un flagello riconosciuto anche nel mondo povero. A tutto questo si continuano ad opporre invece la retorica e una pratica di eradicazione forzata delle colture e credo che tutto ciò verrà confermato a marzo, alla Commissione stupefacenti dell'ONU a Vienna, mentre invece si potrebbero utilmente convertire sia gli sforzi militari, sia quelle colture su altri fronti.

impegnare quattro militari per il mantenimento del cessate il fuoco nella parte nord di Cipro (di cui io sono cittadino) non credo apporti alcunché allo *status* del del nostro Paese all'interno della comunità internazionale. Non che quei quattro militari, se dirottati sul Libano o sull'Afghanistan, possano fare la differenza, ma sicuramente può fare la differenza affrontare la questione nella

Non si può sostenere in quest'Aula che vi è stato un errore amministrativo se ci sono quattro militari a Cipro, perché si dice il falso. Non solo, ma è a verbale dei lavori della Commissione la risposta nella quale c'è scritto che «i limitati contingenti da noi impiegati in alcune missioni, da Haiti al Congo, a Cipro, non vanno considerati come indice di dispersione, ma quale concreta disponibilità dell'Italia a dare un contributo in tutte le principali aree di crisi, secondo gli accordi multilaterali di organizzazioni di cui noi facciamo parte».

Se questo non basta, il Governo è addolorato, ma si domanda: come può convincere il senatore Perduca a non dire falsità in Aula? Posso portare la fotocopia di questo documento, ma basterebbe comunque che si consultasse il resoconto delle sedute della Commissione esteri;

il Parlamento italiano è stato chiamato per ben ventuno volte a votare la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Un dato, questo, che da solo dimostra ormai come si ponga con forza la necessità di mettere mano ad una ridefinizione dell'*iter* legislativo del finanziamento delle missioni Questa esigenza è avvalorata dalla constatazione che ormai ogni sei mesi votiamo dei provvedimenti legislativi che contengono spesso nulla più che singole autorizzazioni di spesa e la riproposizione di disposizioni transitorie relative al trattamento del Il problema non è solo e non tanto la ripetitività della procedura di rifinanziamento. Il punto è che la discussione in Parlamento sta sempre più incentrandosi su aspetti tutto mentre quello di cui si avverte la necessità è che il Parlamento possa incidere in maniera più efficace sulle decisioni relative alle missioni internazionali. Nella realtà odierna, invece (come ha già denunciato il senatore Marcenaro), accade che apprendiamo da un'intervista radiofonica del ministro La Russa di un non meglio precisato aggravarsi della situazione in Afghanistan.

trattazione alla Camera del decreto in titolo, il Presidente della Commissione difesa ha ipotizzato una proposta di esame parlamentare delle missioni internazionali analoga a quella introdotta in materia di finanza pubblica con il DPEF. Ma la riflessione è iniziata nella XIII legislatura con la mozione Rufino. Nella legislatura precedente si è tentata nuovamente una razionalizzazione di questa materia attraverso varie proposte di legge, il cui *iter* è stato interrotto dalla fine anticipata della legislatura. Nei primi mesi di questa legislatura abbiamo ripresentato, come Gruppo PD, nei due rami del Parlamento, specifiche proposte di legge che riprendono quella presentata dalla senatrice Pinotti alla Camera. Credo che siano ormai politicamente maturi i tempi per colmare questo vuoto normativo rispetto alla procedura da seguire in ordine alla deliberazione e all'autorizzazione delle missioni internazionali. internazionali. Altri colleghi sono intervenuti nel dettaglio dell'ammontare dei finanziamenti, dimostrando come sia non vero che, con questo provvedimento, si sia in presenza di un incremento di risorse. In verità, il comparto difesa sta incontrando seri problemi causati dalle scelte operate da questo governo con il decreto legge n. 112 del 2008. Nel mio intervento, per ovvi motivi di tempo, mi riferirò ai problemi relativi alle missioni internazionali che le scelte governative hanno originato. È a tutti noto, infatti, come con il provvedimento in esame vengano finanziati quelli che sono i cosiddetti costi vivi e diretti e che per la copertura complessiva delle missioni internazionali si debba far ricorso al bilancio ordinario della Difesa. Per fare un esempio, le spese per le trasferte del personale vengono finanziate da questo decreto legge fino al 90 per cento. Il vero problema è che, come ci è stato ricordato dai vertici delle nostre Forze armate nel corso delle audizioni, se abbiamo 8.500 unità impegnate in operazioni all'estero, allora dobbiamo tener conto che il numero delle unità coinvolte è almeno il triplo. Questo è dovuto al fatto che tali e tanti sono i militari impegnati nelle varie fasi di approntamento, di recupero, di riorganizzazione al ritorno dallo schieramento operativo. Per non parlare poi di quella che è la struttura logistica, scolastico-addestrativa ed amministrativa che è la base su cui poggia tutta la componente operativa. È questa la struttura che rende materialmente possibile sia la condotta delle operazioni, sia la preparazione delle forze destinate a proseguire nel tempo le stesse operazioni. Un meccanismo estremamente complesso e delicato il cui mantenimento può avere problemi se non adeguatamente finanziato, per quanto attiene sia al reclutamento di nuove giovani leve sia al reperimento di risorse economiche necessarie a garantire il loro addestramento, la manutenzione dei mezzi e il progressivo rinnovo degli equipaggiamenti. Siamo in presenza di un impegno serio, per non dire pesante. E non solo finanziariamente. Uno sforzo finanziario necessario per onorare l'impegno, la responsabilità assunta dall'Italia nel contesto internazionale. Da parte nostra confermiamo il sostegno che abbiamo votato sia quando eravamo al Governo, sia quando eravamo, come oggi, all'opposizione. Un atteggiamento coerente che ci deriva da due valutazioni. La prima è che, per dirla con le parole dell'allora Ministro della difesa, onorevole Arturo Parisi, «quando un Paese assume una decisione, quando formalizza un impegno, ne deriva che la capacità di portare a termine tale impegno nel corso del tempo rappresenta una condizione essenziale perché tale Paese possa essere considerato affidabile, e quindi fattore di stabilità nelle relazioni internazionali». La seconda valutazione è che le missioni internazionali sono parte di una politica estera che si è dovuta e si deve misurare con sfide difficili. Un impegno che ci vede presenti con operazioni NATO su mandato dell'ONU (come nel Kosovo); in missioni di pace dell'ONU (ISAF, UNIFIL); in missioni promosse dall'Unione europea. Sono queste missioni coerenti con il dettato costituzionale che impone all'Italia i vincoli che ci derivano dalla nostra adesione agli organismi internazionali. Esse sono coerenti anche con la necessità di una forte assunzione di responsabilità, da cui dipende anche l'efficacia di una politica multilaterale che, se non produce pace e sicurezza, non serve a nulla. Esse sono la garanzia della difesa degli interessi nazionali, in quanto la stabilizzazione di aree pur apparentemente remote geograficamente

(purtroppo divenute per tutti noi tristemente familiari) è strategicamente centrale proprio a causa della portata globale dei fenomeni destabilizzanti che in tali ambiti trovano la loro origine. La nostra presenza, in Afghanistan, in Libano e nel Kosovo, è molto importante, tanto che ciò ha determinato l'attribuzione al nostro Paese di responsabilità di comando a rotazione con gli altri principali *partner*. sono presenti ed assistono ai nostri lavori, in occasione della loro visita al Senato, gli studenti dell'istituto tecnico commerciale "Federico II" di Capua. A loro e ai loro insegnanti rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività scolastica.

Commissione. Il provvedimento in esame contiene tre elementi nuovi ed importanti che noi della Lega Nord intendiamo sottolineare.

In secondo luogo, si è tornati a prevedere una scadenza semestrale, dopo l'esperienza dei rinnovi di anno in anno, prevedendo una copertura che vede

La terza novità è rappresentata dall'entità delle risorse destinate. Colleghi, parliamo di 808 milioni di euro.

I nostri soldati di pace saranno presenti in tre continenti, dall'Afghanistan al Sudan.

Siamo presenti in tutte le principali aree di crisi del mondo, sparse su tre continenti, l'Asia, l'Africa e l'Europa. Sono 19 le missioni condotte in 22 Paesi. L'Afghanistan, il Libano ed il Kosovo rappresentano sempre il grosso del nostro impegno e dell'impegno delle nostre Forze armate, che in queste tre regioni dislocano l'80 per cento delle risorse messe a disposizione. Non dobbiamo dimenticare missioni meno numerose ma non per questo meno significative. Ricordo, ad esempio, la presenza di 51 finanzieri con finalità di contrasto ai flussi migratori irregolari orientati dalla Libia verso il nostro Paese. Lodevole è anche la nuova iniziativa in Darfur a fianco delle Nazioni Unite e dell'Unione africana. Inevitabile, anche se purtroppo inaspettato, lo sforzo condotto contro la pirateria somala; in questo caso i nostri militari potranno catturare e perseguire in modo adeguato quelli che abbiamo definito i pirati del 2000. Quanto all'Afghanistan, vi sarà un incremento del nostro impegno in quest'area, nella quale il nostro contingente potrà risultare anche più consistente. Un problema da affrontare in futuro e da risolvere - non vogliamo nasconderci dietro alcuna foglia di rosmarino - sarà rappresentato dalla copertura che dovrà essere individuata, in quanto il fondo utilizzato per coprire gli oltre 800 milioni di euro è

L'articolo 2 è dedicato genericamente agli interventi di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione; gli articoli 4 e 5 concedono l'indennità spettante al personale in missione e il regime penale applicabile; l'articolo 6 contiene disposizioni di natura contabile; l'articolo 7 contiene le coperture, e di questo si è già detto; l'articolo 8 dispone infine la consueta procedura accelerata di entrata in vigore. Missione dopo missione il nostro Paese sta dimostrando con i fatti, non con le parole, di stare dappertutto e di contribuire con grande generosità agli impegni internazionali. Non solo, vengono riconosciute perfino dagli amici americani l'attitudine e la capacità dei nostri militari nel ruolo tutto particolare che le varie missioni impongono. Gli amici americani parlano giustamente, e non a caso, di via italiana al *peace keeping*, ossia al mantenimento della pace. Questa via italiana evidenza un mix di capacità militare e di umana comprensione, quindi una ricerca volta più a ciò che unisce I militari italiani hanno comunicato rispetto ed umanità; non sono stati quindi solo valorosi combattenti in Iraq e in Afghanistan, ma anche costruttori di scuole ed ospedali, in tante regioni dell'Africa e dell'Asia, di ponti, di strade e perfino di aeroporti. Non abbiamo occupato nulla nel mondo, abbiamo solo dato: dato: che sia chiaro questo. Il ministro Frattini ben fa a sottolinearlo; il ministro La Russa ben fa ad evidenziarlo, sottolineando quanto è grande la generosità del nostro Paese.

siamo attori principali nella lotta al fanatismo religioso e all'illegalità, oltre che attori principali quanto a generosità e solidarietà.

si viva una crisi internazionale di dimensioni devastanti, nonostante i conti pubblici siano in sofferenza e nonostante i cittadini facciano fatica a

c'era una sorta di commistione tra i fondi utilizzati per le missioni e, soprattutto per la Georgia; i fondi della cooperazione,

il rischio di trovarci ogni volta in una situazione di proroga e per lo più con decretazione d'urgenza, che non permette di affrontare fino in fondo i problemi che riguardano le missioni. Mi riferisco a tre questioni in particolare. So che, soprattutto per conoscenza diretta, anche il sottosegretario Mantica conosce bene queste questioni riferite agli esteri. In primo luogo, essendo ottemperate le ragioni della nostra partecipazione a queste missioni, riguardo ai rapporti con le Nazioni Unite e l'Unione europea, credo che sia arrivato anche il momento di aver un maggiore chiarimento proprio per i dati che anche il collega Filippi ricordava adesso e che la

in Afghanistan c'è una nuova scelta, anche da parte della Presidenza degli Stati Uniti d'America con Obama, che non sarà indifferente rispetto alle scelte che noi dovremo fare anche in quel teatro e in Libano, come abbiamo visto, c'era moltissimo collegamento alle questioni che hanno toccato la striscia di Gaza. In breve, per rimanere assolutamente nei tempi, faccio una riflessione e contemporaneamente rivolgo anche una domanda al Governo in una forma che credo sia costruttiva, anche se proviene dall'opposizione. Non è pensabile che una parte di queste nostre forze impegnate in missioni che sempre più definiamo di pace - non vorrei usare eufemismi - e che svolgono ruoli di controllo internazionale

di truppe alle Nazioni Unite, in seguito agli articoli 43 e 44 dello Statuto ONU, ci permetterebbe in base ad un comma dell'articolo 44 di partecipare anche alle decisioni del Consiglio di sicurezza, in quanto direttamente interessati, anche quando non vi facessimo parte per la forma temporanea.

Credo che la presidenza Obama, che il modello utilizzato da Sarkozy alla Presidenza dell'Unione europea e lo stesso cambiamento dei trattati di Lisbona sulla durata della Presidenza europea portata a due anni e mezzo, proporranno una riflessione che abbiamo affrontato nel nostro Paese solamente ai tempi del Libro bianco di Spadolini o quando si è fatta la riduzione e poi Certo, da Valmy sono passati moltissimi anni, ma credo che una riflessione sul rapporto tra la missione delle nostre Forze armate, soprattutto per la pace,

che sono di fronte a noi, perché si tratta delle missioni militari internazionali di pace e, quindi, del sostegno ai soldati italiani che in queste sono impegnate; in secondo luogo, per la dignità del Senato visto

problematiche principali: un maggior coinvolgimento del Parlamento nell'attività di indirizzo delle missioni all'estero;

un passo in avanti rispetto alla tradizione è già stato fatto con il rinnovo delle missioni

è coinvolto ogni volta che richieda l'intervento del Governo per illustrazioni, dibattiti o discussioni nel merito o nella forma delle nostre missioni all'estero.

piacevoli e costruttivi. Questo per dire che il coinvolgimento della popolazione afgana è la prima ragione della nostra presenza

Gli interventi sono stati profondi, hanno dimostrato un interesse diffuso e - mi sia permesso di dire - anche un'ottima preparazione di tutti.

nessuno ha fatto il minimo riferimento all'entità della copertura o dei costi, ma tutti hanno affrontato il discorso politico. Quindi è giusto - e mi ha confortato quanto detto da Mantica prima - prevedere che il Parlamento possa prima riportarsi ad un discorso politico; quello che tra l'altro -come qualcuno ha ricordato - gli compete. Entro nel merito di qualche particolare considerazione che ha attratto la mia attenzione: mi rivolgo al senatore

di quattro finanzieri di un certo livello che preparano le impostazioni della politica fiscale dell'Albania,

200? Vorrei fare una battuta, sperando che lei non si arrabbi. Per esempio, lei è uno in questo Parlamento; però è efficace: interviene spesso, si fa sentire. Svolge una funzione importante: uno su più di 300. Che vuol dire

È stato posto l'accento sull'opportunità di intervenire fattivamente sulla disattivazione degli ordigni, sulla bonifica di determinate aree, attività che è già in corso: chiunque abbia seguito l'azione dei nostri uomini o abbia avuto la ventura di andare ovunque, in Libano, Afghanistan o in Iraq, ha sentito del loro impegno in tal senso. Trovo giusto che si ponga l'accento su tale aspetto, però il discorso deve essere risolto nell'ambito delle risorse già destinate. Si parla qui di un milione di euro in più, ma chiaramente non è questo il momento per

C'è poi chi ha proposto di prendere già in considerazione la proposta di una copertura per una missione a Gaza; anche questa, secondo me, può essere una dimostrazione di consenso, nell'eventualità però che si dovesse prospettare. È quindi un discorso che mi sembra anticipato. Certo, vi è

di un attento monitoraggio delle aree in cui vengono impiegati nostri militari o civili ed anche le organizzazioni non governative, che generosamente si prodigano per prevenire eventuali conseguenze negative

Chiedo al Governo se può accogliere come raccomandazione

perché corrispondeva allo spirito e alla sostanza delle esigenze che anche noi avevamo prospettato. Per queste ragioni ritiro l'emendamento 3.4, di cui sono il primo firmatario, che riguarda

sono state fatte presenti già in sede di discussione alla Camera le perplessità del Governo relativamente alla parte del dispositivo testé richiamata dal rappresentante del Governo, tolto quanto letto dal sottosegretario Mantica, il testo possa essere considerato accettabile e quindi accolto come raccomandazione. Siccome abbiamo una pausa di tre ore per riformulare eventualmente il dispositivo, se ci fosse la disponibilità a prendere in considerazione una riformulazione magari proprio cancellando quelle due righe, credo che in effetti si darebbe il segnale, che si auspicava poco fa durante la discussione generale, di avere una legge sotto la quale tutti siamo da trattare nello stesso modo.

senatore Ramponi è d'accordo?

Prego, senatore. si sono verificati numerosi e gravi infortuni sul lavoro. In particolare voglio ricordare che il 13 febbraio a Brescia è morto un operaio albanese, precipitato da un tetto; nella stessa giornata a Gaiole in Chianti un uomo di 79 anni è morto schiacciato dal trattore; il 14 febbraio a Campo nell'Elba, in Provincia di Livorno, un operaio è morto lavorando in un cantiere edile; il 16 e il 17 febbraio ci sono stati altri tre infortuni mortali in provincia di Savona, di Ascoli Piceno e di Gorizia. Quindi, credo anch'io - come la settimana scorsa dal senatore Nerozzi - che sia necessario, davanti a tragedie di questa entità che non tendono a contenersi, che il Governo venga a riferire su come sta operando in termini di attuazione del Testo unico. In particolare, penso che il ministro Sacconi

per fatto personale circa le accuse di aver mentito che mi sono state rivolte da parte del rappresentante del Governo che naturalmente, come tutto il Gruppo del Popolo senatore segretario Malan, non è in Aulain questa fase dei lavori. Un conto è dire che una persona non ha risposto, cosa che io non ho fatto relativamente a quanto è stato detto dal Governo in sede di dibattito in Commissione, altro conto è dire che le argomentazioni che sono state portate a spiegazione di determinati tipi di scelte sono del tutto risibili. Ci sono quattro Carabinieri disarmati che mantengono un cessate il fuoco a Cipro nord. Invito il sottosegretario Mantica a recarsi a Cipro nord e poi mi saprà dire se c'è bisogno di tenere sotto

che ha già interamente distrutto una palazzina del centro. Le operazioni di spegnimento del rogo sono rese difficili oltre che dal forte vento, anche dai pochi mezzi a disposizione, anche perché l'unico presidio dei Vigili del fuoco è all'interno dell'aeroporto. Altre agenzie informano che le fiamme all'interno di questo campo erano alte dieci metri e che è stato distrutto uno dei tre blocchi, dove vivono 900 persone invece delle 300 previste. notte, con la speranza che non ci sia rimasto qualcuno dentro mentre divampava l'incendio e che non piova, 300-350 persone dormiranno all'addiaccio in un centro che nel giro di tre giorni è stato trasformato da centro di prima assistenza e soccorso in CIE vero e proprio.

Signor Presidente, qualche giorno fa il Ministro dell'economia francese Christine Lagarde ha diffidato i banchieri che ricevono aiuti pubblici dall'incassare *stock option*, prebende e perfino i dividendi. In Italia, invece, è stato approvato un decreto che dà aiuti pubblici ai banchieri privati. ci sono tre banchieri privati che hanno guadagnato, nel 2007, circa 25 milioni di euro, il controvalore di 2.500 precari. Questi banchieri rispondono al nome di Gabriele Galateri,

alla questione, non personale, ma relativa al Centro di identificazione ed espulsione di Lampedusa, che ha sollevato il senatore Perduca, chiederò al presidente Schifani di valutare

ci auguriamo tutti ed esprimiamo l'auspicio che la situazione sia controllata e che non si creino disagi e rischi per la vita delle persone e degli operatori dei Vigili del fuoco impegnati ad affrontare una situazione, che da già difficile rischia di diventare ancora più drammatica.